Signor Presidente, prego lei e gli onorevoli colleghi di dedicarmi appena un attimo di attenzione sull'ordine dei lavori o, meglio, sull'apertura dei nostri lavori.

che impegnano una Camera del Parlamento. Ma ancora ieri e anche questa mattina registriamo una sorta di delegittimazione diffusa della nostra affidabilità, dei nostri lavori e delle nostre persone nella stampa e anche nel gran parlare che ciascuno di noi affronta nelle proprie città e nei propri luoghi di frequentazione riguardo alla presunta dilagante diffusione di droghe e stupefacenti di ogni genere tra i parlamentari. Vediamo anche arrivarci messaggi, segnalazioni o inviti a decidere se sottoporci o meno ai relativi test di verifica. signor Presidente, vorrei affidarle una breve considerazione e anche una richiesta. La considerazione è che,

esiste ancora la raccolta differenziata e che il costo di tale raccolta è legato non tanto alla quantità

nato dall'esigenza di affrontare complessivamente il problema della finanza pubblica non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale e di

che il Governo ha inserito nel programma e che vuole portare avanti. Anche in questo caso, a causa dei vincoli di bilancio, non possiamo definire complessivamente il tema, però è sicuramente uno degli obiettivi della scelta politica complessiva del Governo che verranno comunque perseguiti.

che si intervenga aumentando le detrazioni, in particolare sui redditi da lavoro, cercando in questo modo di operare un intervento che vada sia nella direzione di una maggiore equità sociale e di un recupero della capacità reddituale dei redditi da lavoro, che negli ultimi dieci anni hanno perso moltissimo potere di acquisto, sia nella direzione di una spinta alla ripresa dei consumi come stimolo indispensabile per avviare il percorso di uscita dalla crisi nel nostro Paese. Questa finanziaria non si sta occupando del lavoro e dei redditi da lavoro e da pensione, e a noi questo sembra gravissimo in un momento in cui

francamente che sono molto stupito del fatto che sia il relatore di maggioranza che il Governo non abbiano degnato questo emendamento di una qualche considerazione. In buona sostanza, signor Presidente, si tratta di quanto Il Governo, nel corso di questo anno e mezzo, ha sviluppato un solo intervento significativo in termini di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. È l'intervento - uno dei primi assunti dal Governo di centrodestra subito dopo la sua costituzione - relativo alla detassazione della quota di salario da lavoro straordinario e alla detassazione della quota di salario da contrattazione di secondo livello. Sulla prima parte di questo intervento, la crisi è intervenuta mettendolo sostanzialmente in non cale. Il Governo ha approvato un provvedimento a favore della riduzione della pressione fiscale sugli straordinari; nel frattempo sono scomparsi gli straordinari, per cui il problema è stato "risolto" alla radice. Ma non c'è dubbio che, dal punto di vista qualitativo, la seconda parte di questo intervento, cioè la detassazione della quota di salario da contrattazione di secondo livello, era una scelta che il Governo giustamente - a mio avviso - ha presentato come strategica. La riduzione della pressione fiscale sulla quota di salario da contrattazione di secondo livello è infatti una scelta che tende, da un lato, ad affrontare la questione salariale, dall'altro, ad affrontarla nel senso che si premia quel rapporto tra le parti volto innanzitutto a misurare consensualmente la crescita della produttività e, secondariamente, a premiarla attraverso un aumento del salario su cui peraltro lo Stato, al fine di sviluppare la contrattazione di secondo livello, interviene fiscalmente per favorirla. Il fatto incredibile è che quella scelta qualitativa, e positiva, del Governo di centrodestra con la finanziaria di quest'anno viene completamente definanziata. Nelle audizioni, le parti sociali - da Confindustria alle organizzazioni sindacali - ci hanno chiesto qual è la logica in base alla quale anche l'unico intervento che è stato fatto viene definanziato con la finanziaria. Noi proponiamo un emendamento che è volto a prevedere le risorse per per continuare almeno a fare quanto si è fatto nello scorso anno per finanziare la detassazione della quota di salario da contrattazione. Sarebbe stato ragionevole seguire l'indicazione che ci hanno dato alcune organizzazioni sindacali e datoriali, le premiare lo *start-up*, cioè la scelta di fare contrattazione di secondo livello là dove non si fa ancora; pertanto c'è bisogno di concludere il primo accordo in questo senso. Invece di premiare l'inizio della contrattazione di secondo livello anche dove non si fa, il Governo inopinatamente definanzia quel poco di positivo che aveva fatto. C'è da restare allibiti: non siete nemmeno capaci di dire una parola su questo argomento! Trovo davvero che ci sia da rimanere esterrefatti per la pochezza con cui state contornando il nulla di questa legge finanziaria!

indica un primo intervento di detassazione a cominciare dalla tredicesima.

le possibilità di spendere e di alimentare la domanda interna.

anche l'emendamento 2.25 interviene sul tema del potere d'acquisto dei redditi medio bassi, cioè dei redditi da lavoro dipendente e da pensioni. Si tratta di un argomento che da un anno stiamo introducendo in tutte le nostre proposte e nei nostri interventi, perché siamo convinti che l'economia potrebbe ripartire anche dai consumi. Quest'anno abbiamo visto una forte contrazione sia delle esportazioni che dei consumi interni. Ciò ha prodotto una diminuzione della produzione con la conseguente crisi di tantissime aziende: sul potere d'acquisto di quei redditi che maggiormente sono stati erosi in questo periodo, si potrebbe dare, appunto, un forte impulso anche ai consumi. L'emendamento 2.25 agisce sul tema del trattamento pensionistico, intervenendo direttamente sul decreto-legge n. 81 del 2007, convertito nella legge n. 127 del 2007. Si tratta della legge che, in qualche modo, istituiva la cosiddetta quattordicesima mensilità per le pensioni. Con l'emendamento proposto si provvede, attraverso diverse modalità contenute anche nella tabella presentata, in due modi: ampliando la platea dei beneficiari di queste misure incrementando le somme da erogare. Per la copertura noi proponiamo alcuni tagli sulla spesa pubblica. Il Governo finora è stato assolutamente sordo rispetto a questo tema. Noi auspichiamo che vi sia un cambio di rotta perché, in questo modo, si potrebbe dare una risposta a tutte quelle famiglie che sempre più stanno vivendo in condizioni disagiate e stanno guardando con grande preoccupazione al proprio futuro.

Riteniamo insoddisfacenti gli interventi che il Governo ha sinora attuato in questo senso: il fondo di garanzia spesso è stato solo al servizio della grande impresa applicato l'avviso comune, sottoscritto nei mesi scorsi tra il Governo, l'ABI, il sistema bancario e le organizzazioni delle imprese nel nostro Paese, per una moratoria dei mutui e delle operazioni di finanziamento a cui le imprese hanno attinto negli anni passati.

Presidente, intendo richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi della maggioranza su questo emendamento, che si propone di sostenere le imprese che operano sui beni confiscati alle organizzazioni mafiose rendendo loro accessibile il Fondo per la gestione separata della Cassa depositi e prestiti. Lo scorso venerdì pomeriggio a Bologna il ministro Maroni ha vantato gli importanti risultati raggiunti dal Governo nella confisca dei beni alle organizzazioni mafiose, sostenendo che in un anno e mezzo sono stati sequestrati 5.000 beni. Questo è senz'altro un risultato importante, che rischia però di essere totalmente vanificato se questi beni non possono essere gestiti con risorse adeguate dagli enti locali e dalle organizzazioni e imprese sociali a cui vengono affidati in forza della legge n. 109 del 1996. Si tratta quasi sempre di piccole imprese che ad oggi hanno

nel riconoscere che l'acqua è una risorsa strategica non solo per il settore dell'agricoltura ma per l'intero Paese. È altrettanto vero che a fronte delle dimensioni di una eventuale ristrutturazione e contingentamento delle acque nel nostro Paese una sola legge finanziaria non basta. Ciò che manca, però, a questo Governo e a questa maggioranza è la capacità di fare propria la cultura della manutenzione del territorio. Ciò che non fa effetto non interessa e, quindi, siccome interventi programmati nel tempo hanno poca possibilità di essere percepiti e individuati non vengono

affermare che l'agricoltura è stata fortemente penalizzata, anzi direi totalmente ignorata da questa finanziaria ed è per questo che il Partito Democratico ha presentato una serie di emendamenti e di ordini del giorno su alcuni punti strategici, proprio per recuperare le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza. Mi riferisco, in particolare, agli emendamenti e agli ordini del giorno volti a recuperare risorse per la previdenza, per stabilizzare il regime di agevolazione contributiva in agricoltura nelle zone svantaggiate e nelle zone di montagna, che scade il 31 dicembre, la cui sospensione metterebbe in ginocchio l'intero sistema agroalimentare del Paese, in particolare delle zone del Mezzogiorno. Mi riferisco al fondo di solidarietà nazionale, al credito di imposta sugli investimenti relativi a macchinari e attrezzature agricole, all'accesso al credito e alla rinegoziazione dei tempi. Penso che siamo di fronte ad una emergenza e che l'emergenza vada affrontata con provvedimenti tempestivi e di immediata efficacia: sarebbe inutile intervenire con la cura quando la malattia è giunta ad una fase irreversibile, terminale. Occorrono, quindi, da un lato interventi immediati per garantire il sostegno minimo necessario per arginare la crisi; dall'altro politiche di lungo respiro per promuovere lo sviluppo e la competitività. In tale contesto è da registrare purtroppo, ancora una volta, l'assenza di risposte

Avete detto di no anche ai corsi di lingua e cultura per i discendenti di italiani all'estero; avete detto di no anche a quattro spiccioli per i cittadini italiani nati in Italia che vivono in Sud‑America in stato di indigenza, però continuate a dire di sì ai miliardi puliti puliti che gli italiani all'estero fanno rientrare in Italia (non quelli sporchi dello scudo). Allora pregherei di rispettare un attimo di silenzio alla memoria delle prime righe dell'articolo 3 della nostra Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità

recuperare un po' di risorse rispetto ai tagli triennali previsti dalla legge n. 133 del 2008. Stamattina in diretta il ministro Gelmini ha detto che l'università è strategica e importantissima per questo Paese.

È stato presentato il disegno di legge sull'università, che non è finanziato e si parla di finanziarlo con lo scudo fiscale. Eppure, dal momento che i tagli sono triennali, prevedete forse tre scudi fiscali consecutivi? Vi chiediamo di appoggiare questo emendamento che reintegra parte delle risorse.

le spese relative all'acquisto dei testi scolastici per le famiglie italiane; credo sarebbe un buon segnale, considerato che in questa finanziaria, allo stato, per la famiglia c'è poco o nulla: meglio, c'è il nulla!

Signor Presidente, vorrei ricordare ai nostri colleghi che se c'è un investimento vero che possono fare le famiglie è l'investimento sugli studi a tutti i livelli, per arrivare alla massima capacità di partecipare al progresso ed allo sviluppo del Paese. Le classi medio-basse sono quelle che in questo momento rischiano di non avere lo stipendio; figurarsi se hanno i libri di testo! Quindi, chiediamo al Governo di detassare i libri di testo, dalle scuole superiori all'università. Ci sembra sia una misura minima per aiutare le famiglie, visto che continuiamo a parlare di aiutare le famiglie a partire dal quoziente familiare.

abbiamo approvato assieme, quindi con voto *bipartisan,* una mozione proprio su questo (il Presidente mi sta appunto dicendo di sì con la testa).

dalla collega Garavaglia, e che nella mozione a mia prima firma avevamo presentato, era proprio quella di sgravare le famiglie da questa spesa che sta diventando sempre più onerosa, finalità sulla quale il Governo aveva dato il suo parere. Credo che incentivare la cultura

cogliamo l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Aula su questo emendamento, che consideriamo un piccolo ma importante segnale che il Governo potrebbe dare alle famiglie italiane.

il Parlamento europeo ha approvato nei primi mesi di quest'anno una risoluzione con cui si chiede agli Stati membri la possibilità di esaminare con attenzione l'applicazione dell'IVA agevolata sui prodotti dell'infanzia, proprio per favorire non solo una politica a sostegno delle famiglie ma,

caso l'IVA agevolata significa poter dare un sostegno indiretto a tali famiglie, in quanto diversi dati economici ci fanno ritenere che

Vedete, questa è una proposta che considero, usando un termine di questi tempi, *bipartisan*, perché al riguardo già diversi sindaci ed amministratori del centrodestra si stanno muovendo. tra gli ultimi anche il sindaco di Roma, il quale ha sottoscritto un'intesa con il sindaco di Madrid proprio per promuovere una petizione europea

di dare questo piccolo segnale a sostegno delle famiglie, soprattutto di quelle che hanno un grave disagio sociale, applicando l'IVA agevolata che già esiste in diversi Paesi, che forse hanno più deficit di noi

meno tasse e più sicurezza. Sul più sicurezza, con le relative risorse economiche, bisogna rivolgere la domanda alle forze dell'ordine, che stanno protestando in questi giorni, e al ministro Maroni, che protesta con il Ministro dell'economia. Sul meno tasse bisogna chiedere ai 28 milioni di italiani che pagano onestamente le tasse rispetto a chi usufruirà dello scudo fiscale. Almeno, noi chiediamo a questo Parlamento un piccolo segnale applicando quella misura di IVA agevolata, che altri Paesi europei, forse più civili del nostro, hanno già applicato.

È vero che sull'istituto del 5 per mille ampio e vasto è il consenso e che si sta lavorando di concerto fra maggioranza e opposizione per definire un provvedimento che lo stabilizzi, in modo da farci evitare ogni anno il solito tormentone di trovare la garanzia e la copertura finanziaria.

Chi conosce il mondo del volontariato sa che una delle domande che viene rivolta è quella di avere certezza sulla possibilità di pianificare e programmare le proprie attività, che già risentono della circostanza che le persone vi

si parli tanto nei convegni ma che poi, all'atto pratico, se ne neghino i presupposti e le condizioni di sostegno e di operatività.

Come mi è capitato di richiamare in dettaglio in discussione generale, sono oltre tre i miliardi in riduzione sulle infrastrutture rispetto al consolidato 2009 e sono quasi 400 milioni di euro sul programma di sviluppo della mobilità locale, di cui 124 milioni a riduzione delle risorse disponibili per il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale, 100 milioni per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale, 50 milioni per elevare il loro livello di sicurezza, 56 milioni per realizzare il trasporto rapido di massa e tranvie e 48 milioni per favorire la realizzazione dei sistemi ferroviari passanti. Da queste cifre è fin troppo facile prevedere i disagi e le sofferenze che verranno scaricati sui lavoratori delle aziende di trasporto e sugli enti locali e le Regioni, titolari di questi servizi a vario titolo, in prima linea nel far fronte alla quadratura dei conti per l'equilibrio dei bilanci e al contempo il mantenimento di servizi sempre più onerosi, per effetto delle fluttuazioni dei costi energetici e degli incrementi inflattivi più generali. Con questo emendamento, onorevoli colleghi, chiediamo che per questi inevitabili disagi che saranno prodotti siano almeno parzialmente risarciti i cittadini e le imprese, gli utenti di questi servizi, consentendo loro sgravi fiscali in detrazione dall'imponibile IRPEF - e IRAP per le imprese - per i titoli di viaggio e per gli abbonamenti dei lavoratori pendolari e degli studenti. Tra l'altro, trasferire quote crescenti di passeggeri dal trasporto privato, spesso individuale, al trasporto pubblico collettivo costituisce o dovrebbe costituire sempre più l'azione di intervento principale a favore dello sviluppo di una mobilità sostenibile secondo gli Accordi di Kyoto, che per il nostro Paese prevedono proprio nella riconversione dei mezzi di trasporto e in un riequilibrio della mobilità a favore dei servizi pubblici collettivi come si dice in gergo, dalla gomma alla rotaia - la principale azione di intervento per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'aria. Voteremo quindi convintamente a favore di questo emendamento, ma riteniamo sarebbe anche apprezzato dai cittadini un vostro appoggio in tal senso.

l'Italia arriva a questo appuntamento senza avere le carte in regola, senza aver cioè rispettato quegli accordi, dei quali pure siamo stati protagonisti nel G8 dell'Aquila, che prevedevano un impegno importante dei Paesi sviluppati a favore dei Paesi più poveri, e che, soprattutto, consideravano quest'impegno non come un aspetto contingente e assistenziale ma come parte strutturale

la lotta alle pandemie e, in particolare, il finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi. Si tratta di malattie in espansione, mentre esistono tutte le possibilità

questa responsabilità è, a nostro avviso, una scelta ineludibile da parte del Governo italiano come di quelli degli altri Paesi più sviluppati.

che questi finanziamenti prevedono anche un sostegno particolare per la creazione di nuove imprese femminili e per il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili. In questo periodo di crisi non è certo con la cassa integrazione che si danno risposte, ma con

Ristrutturare una casa è decisione che richiede un po' tempo per ottenere i preventivi e le autorizzazioni, dove previste. È evidente che da oggi in poi regnerà l'incertezza, e che l'efficacia che questo strumento ha avuto fino ad oggi - ricordo che grazie all'incentivo sono stati aperti quasi

che ne beneficiano, le famiglie, sostanzialmente cesserà. Questa è la ragione per cui torniamo a chiedere con forza il rifinanziamento dell'incentivo del 55 alle ristrutturazioni energetiche, sperando che il Governo e la maggioranza ci dicano almeno che non sono d'accordo, oppure, se sono d'accordo, che mostrino poi una qualche coerenza e conseguenza.

alle proposte e agli indirizzi del Governo nazionale sull'istituzione della zona franca nelle aree colpite dalla grave tragedia del terremoto.

anche perché, in considerazione del fatto che l'Unione europea ha approvato proprio di recente l'istituzione di 22 zone franche, di cui una in Abruzzo, però nella fascia nella fascia costiera della nostra Regione, c'è la necessità, per rilanciare effettivamente l'economia di questi territori martoriati, di dare adeguata copertura economica e immediata prontezza

e che voi, invece, con i provvedimenti assunti nel corso di questo anno e mezzo, avete demolito pezzo per pezzo. Il nostro Paese sta così vivendo un imbarazzante paradosso: mentre questa crisi richiama tutti noi, a livello internazionale, a perseguire la strada di una finanza fondata sul rispetto delle regole e della trasparenza; mentre questa crisi ci richiama al tema della legalità quale presidio di coesione sociale e di civismo responsabile, qual è la risposta? Si smantellano le norme sulla lotta all'evasione ed elusione fiscale e si approva lo scudo fiscale. Noi chiediamo invece che riacquistino efficacia le disposizioni volte a dar corso con rigore e serietà a quegli strumenti di controllo e di vigilanza che facciano emergere l'economia sommersa e illegale dalle enormi dimensioni che tutti conosciamo. Tutte misure che voi avete cancellato, rinunciando così a percorrere quel cammino progressivo, serio e costante di recupero dell'evasione ed elusione fiscale che avevamo iniziato a tracciare. È un discorso di equità, di giustizia, di rispetto del patto fiscale fra Stato e cittadini, fondato sulla responsabilità e non certo sulla insostenibile sperequazione di cui oggi quel rapporto soffre, ed è, soprattutto in una fase come questa, la strada per recuperare risorse urgenti da destinare alle misure che con gli altri emendamenti illustrati dai colleghi del Partito Democratico abbiamo proposto a favore dei redditi medio-bassi e delle famiglie disagiate, sui quali gli effetti della crisi impattano in modo drammatico. Per questo votiamo convintamente a favore dell'emendamento

che da anni attende un rifinanziamento adeguato e che nelle ultime azioni del Governo è quasi totalmente scomparso, con grave danno, credo, per l'imprenditoria in generale e per quella femminile in particolare.

per l'area del cratere del terremoto, è assolutamente insufficiente, converrà con noi, signor Presidente, che la situazione di crisi industriale nell'area del terremoto è estremamente pesante e che

Chiedo ai senatori Lusi e Legnini la possibilità di aggiungere la firma dei senatori abruzzesi dell'Italia dei Valori,

questa mattina la stampa ha riferito di una presa di posizione dell'Assemblea generale dei vescovi italiani. I vescovi chiedono che si dica la verità, non si prometta l'impossibile creando aspettative e illudendo la gente, che non sono ammissibili giochi mediatici sulla ricostruzione e sul post terremoto. Sempre questa mattina, signor Presidente, onorevoli colleghi, un fisico importante, Gaetano De Luca, ha

i feriti e i dispersi del terremoto del 6 aprile. Morti che stiamo dimenticando - ahinoi! - troppo in fretta, così come stiamo dimenticando che migliaia di famiglie ad oggi, mese di novembre, sono ancora senza una sistemazione, nonostante gli sforzi positivi che sono stati fatti per la costruzione delle case transitorie: sono ancora almeno 6.000-7.000 le famiglie che non hanno una sistemazione. sistemazione. Stiamo dimenticando in fretta che la ricostruzione vera ad oggi non è ancora iniziata: per nessun edificio, né di civile abitazione, né produttivo, né pubblico né con altra destinazione oggi è stata avviata l'attività di ricostruzione. L'emendamento in titolo, signor Presidente, signori della maggioranza, signori del Governo, vuole affermare un principio molto semplice, peraltro poco oneroso, e cioè che coloro che sono deceduti o sono rimasti gravemente infortunati in occasione di quel sisma, che si è determinato anche a causa dell'uomo, siano equiparati agli infortunati del lavoro. È un emendamento che potete e che possiamo approvare; è un emendamento che ci aiuta a non dimenticare e a fare un po' di giustizia.

inserimento di un comma 8*‑bis* trova motivazione nella *ratio* stessa del Fondo di solidarietà nazionale. È uno strumento vitale, di grande importanza per arginare i rischi connessi a qualsiasi attività agricola. un meccanismo di gestione del rischio in agricoltura in grado di potenziare il ruolo delle polizze assicurative attraverso l'adesione in forma collettiva ad uno dei consorzi di difesa oppure ad una cooperativa che esercita l'attività di difesa a favore degli associati. Questa è la ragione per la quale il Gruppo del Partito Democratico ritiene necessario provvedere al rifinanziamento delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale, con 480 milioni di euro per il 2010 e con la retroattività per il pagamento dei saldi contributivi relativi agli anni 2008 e 2009. Siamo in una situazione particolare. Quest'anno, e nel tempo anche molto recente, vi sono state varie fenomenologie e calamità naturali, che purtroppo sono coincise con l'assenza di finanziamento del Fondo, che hanno determinato una strana ricaduta in parecchi casi sul territorio nazionale; gli agricoltori non hanno stipulato polizze assicurative e quindi sono completamente scoperti. È facile ritenere, signor Presidente, che questo emendamento subisca, ahimè, la stessa sorte di tanti altri e che venga bocciato. È ben strano constatare che nel frattempo, durante l'esame alla Camera dei deputati del decreto sulla competitività nel settore agroalimentare (Atto Camera n. 2260), lo scorso il ministro Zaia abbia preannunciato l'introduzione di un articolo 2-*bis*, con il quale si stanziano 122 milioni di euro per il Fondo di solidarietà nazionale e per gli incentivi assicurativi riferiti all'anno 2010, prevedendo così la possibilità di coprire parte del fabbisogno anche degli anni precedenti. Questi 122 milioni di euro sono attinti o sottratti, a seconda di come la si vede, dal fondo per filiera agroenergetica o piuttosto, come ha detto il ministro Zaia, dallo scudo fiscale, come ha affermato alla Camera lunedì scorso. Vorremmo capire la ragione di questo meccanismo a doppia velocità: ciò che si nega al Senato, disattendendo una diffusa quanto legittima aspettativa delle imprese agricole dell'intero territorio nazionale, poi si concede, seppure con un finanziamento più ridotto, presidente Scarpa Bonazza Buora, alla Camera dei deputati. Ci sono altre questioni affrontate dall'emendamento 2.246 che tratto solo per titoli: la proroga annuale del regime di agevolazione contributiva in agricoltura nelle zone svantaggiate e di montagna; montagna; la disciplina dell'istituzione di un fondo per lo sviluppo dei Confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare ed ancora il finanziamento di un fondo a favore dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Si vuole, inoltre, rendere più efficace la disciplina in materia di credito d'imposta

a nome del Gruppo del Partito Democratico, il voto favorevole a questo emendamento.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori esprime la sua più netta contrarietà al contenuto del presente comma 8-*bis*, che si configura, specialmente per quanto concerne il contenuto del secondo periodo dello stesso, come un ennesimo incentivo all'evasione fiscale. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) veniva istituito nel 2002, con la legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di semplificare l'attestazione della regolarità contributiva da

requisito necessario per l'accesso a finanziamenti comunitari. La finanziaria 2007 aveva stabilito di subordinare al possesso del DURC anche la fruizione di benefici normativi e contributivi.

Secondo tale provvedimento chi non risulta in regola con gli adempimenti contributivi non può ottenere l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche o in forma itinerante. inoltre, il DURC diviene condizione necessaria per il rinnovo annuale dell'autorizzazione stessa da parte del Comune competente e, per questo, deve essere ripresentato entro il 31 gennaio di ogni anno. La stessa maggioranza che non più tardi di quattro mesi fa approvava il decreto-legge n. 78 oggi torna inopinatamente sui propri passi. Un ulteriore e più grave aspetto negativo dell'inserimento del comma 8-*bis* emerge dalla lettura del secondo periodo del comma stesso: «Si intendono comunque «Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici nazionali

che fino ad oggi si sono comportati onestamente, ottemperando a tutti gli obblighi di legge, concedendo viceversa quegli stessi vantaggi agli eventuali abusivi. Ci farebbe piacere conoscere - lo chiedo ai colleghi che hanno presentato tale modifica - quale sia stata la causa di questo cambiamento repentino di rotta rispetto al decreto anticrisi, tenuto conto che la stessa Associazione nazionale venditori ambulanti (ANVA) conviene sulla necessità del mantenimento dell'obbligo di presentazione del DURC, proprio al fine di combattere il diffondersi di abusivismo e lavoro irregolare. Invito pertanto tutti i colleghi a votare positivamente la nostra richiesta di sopprimere il secondo periodo del comma 8-*bis*. Chiedo inoltre che

la dichiarazione di voto del Partito Democratico è favorevole a questo emendamento, perché il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione è spesa certa, che non può essere disattesa nella formazione di una legge finanziaria. Consideriamo il raddoppio degli stanziamenti annuali il minimo che il Governo debba mettere a disposizione della contrattazione per i lavoratori, che già devono devono subire provvedimenti che tendono a demonizzare la categoria della pubblica amministrazione, e soprattutto per conservare il potere di acquisto. Non dimentichiamo inoltre che, se da una parte si favoriscono gli evasori fiscali con lo scudo fiscale, dall'altra i lavoratori dipendenti sono i più sicuri e numerosi contribuenti del fisco. E vengono sempre demonizzati.

del ricorso alla cassa integrazione ordinaria del 500 per cento (ossia moltiplicata per cinque volte), una cassa integrazione ordinaria - come si ricava anche dalla lettura dei quotidiani di oggi, in particolare relativamente al caso FIAT, ma non solo - che si sta esaurendo.

il trattamento di disoccupazione, e in particolare che venga esteso ai lavoratori che oggi ne sono sprovvisti. Ricorderete che nei mesi scorsi il Partito Democratico ha presentato una richiesta specifica a tale riguardo chiedendo un assegno di disoccupazione. In secondo luogo, chiediamo l'estensione della cassa integrazione ordinaria a quei lavoratori e lavoratrici, a quelle imprese che oggi non sono assolutamente Ovviamente la risposta non può essere, come è stata finora da parte del Governo, la cassa integrazione in deroga, essendo questa da un lato insufficiente e dall'altro, quando arriva, arrivando in ritardo, lasciando i lavoratori e le lavoratrici interessati scoperti per quanto riguarda il sostegno al In terzo luogo, chiediamo il raddoppio fino a tutto l'anno 2010 della cassa integrazione ordinaria. Si dirà - l'abbiamo già sentito in altre circostanze - o addirittura non si dirà niente da parte da parte del Governo, il che è lo stesso, che non ci sono le risorse. A questo riguardo vorrei ricordare che la Presidenza del Gruppo del Partito Democratico ha presentato nei giorni scorsi una interrogazione specifica, nella quale si dimostra che che il fondo della cassa integrazione ordinaria negli ultimi cinque anni ha registrato un avanzo di circa 12 miliardi di euro. Quindi, non è assolutamente vero che non ci sono Quindi, non è assolutamente vero che non ci sono le risorse. Quello che risulta di tutta evidenza è la volontà politica del Governo di scaricare i costi della grave crisi sociale unicamente sui lavoratori dipendenti, e questo ci sembra particolarmente inaccettabile.

la grave crisi (non psicologica) getta sul lastrico moltissime imprese, soprattutto al Sud. Grandi aziende chiudono, fanno appelli sui giornali per sensibilizzare le istituzioni. Le microimprese, sottocapitalizzate, continuano ad avere nel sistema bancario non certo un alleato. Il contrasto all'usura in questa fase è fondamentale. La morsa del racket continua ad alimentare le casse della mafia e delle altre organizzazioni criminali. Tutto ciò avviene nonostante l'impegno dell'associazionismo antiusura e antiracket, unitamente all'encomiabile opera di poliziotti, carabinieri, finanzieri, che operano senza auto, senza benzina, senza straordinari e senza adeguamento degli stipendi. Il combinato disposto della diminuzione degli stanziamenti per il contrasto all'usura e al racket, unitamente al blocco delle intercettazioni e al fumo negli occhi delle ronde miste, è la vera cartina di tornasole del vostro impegno, che non si compensa ed anzi stride con il numero degli arresti. Ecco perché invito i colleghi a votare questo emendamento per dare una forza in più, per dare dignità a chi denuncia, molto spesso nella paura, sia usura che racket.

per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. Invito i colleghi ad una puntuale riflessione sulla situazione del sistema sicurezza a seguito delle decurtazioni di bilancio registratesi anche quest'anno, che hanno indotto, come giustamente ricordava il collega Pegorer ieri nel suo intervento illustrativo, i sindacati nonché decine di migliaia di operatori e di operatrici delle forze di polizia e delle Forze armate a manifestare lo scorso 28 ottobre nelle PIAZZE della capitale. Tra le conseguenze di queste decurtazioni forse la più preoccupante è la demotivazione che può colpire gli addetti alla sicurezza per la mancanza di strumenti (in particolare di strumenti tecnologici aggiornati) e di strutture funzionali e anche per la mancanza di una visione strategica degli investimenti coerente con la passione e la professionalità che donne e uomini del comparto sicurezza pongono quotidianamente sul fronte delle criminalità mafiose, mietendo successi straordinari. è la demotivazione che può venire agli addetti alla sicurezza per quanto riguarda la prevenzione tecnica. Quest'ultima è un sistema molto vicino al cittadino nei vari contesti territoriali, territoriali, e i suoi risultati non usufruiscono della scenografia mediatica, ma sono invece affidati al dato freddo della statistica, molto spesso strumentalizzata in senso negativo. Questi due emendamenti dovrebbero essere votati all'unanimità per sollecitare il Governo ad adottare, a concertare e a condividere un piano, un progetto, un programma pluriennale per recuperare il per recuperare il senso generale e sistemico di tutto l'apparato dedicato alla sicurezza, anche al fine di evitare che nelle prossime manovre finanziarie venga ulteriormente oltraggiato il sistema stesso. Tutto ciò è fortemente auspicabile non soltanto per restituire decoro, dignità e funzionalità agli operatori del sistema sicurezza, ma anche per rendere meno incredibili - consentitemelo

la questione del 5 per mille, del volontariato, non è di destra o di sinistra, ma riguarda tutti coloro che si prodigano ogni giorno per aiutare i deboli, gli ultimi, la ricerca, le università, i Comuni che si finanziano. Questa mattina

tratta, come è già stato rilevato, dell'arruolamento del personale volontario e del mantenimento in servizio di coloro che stanno operando in tanti teatri di crisi nel mondo.

bensì per diventare un centro di acquisti, un collettore di beni e servizi, per la modica cifra di circa cinque miliardi l'anno. Che cosa si intende fare, signora Presidente? Sono contento di potermi rivolgere a lei. dicevo, sono contento di potermi rivolgere a lei perché questo emendamento non solo si riferisce ad una norma intrusa, intrusa, ma tenta di smascherare una vera e propria espressione di saccheggio dell'ultima normativa vigente, e quindi di quella cogente, relativamente alla formazione della legge finanziaria.

Parlo a beneficio anche del mio collega sardo, senatore Sanna, che solo perché ho parlato di decenza ha voluto urlare ma, visto che siamo nella stessa posizione, non so se si riferisse a me o al sottosegretario Giovanardi.

Forze armate delle quali la maggioranza si riempie la bocca in ogni circostanza e che, oltre ad essere ridotte al lumicino che da 191.000 unità si scende a 120.000), oltre a non poter seguire corsi di addestramento, oltre a dover licenziare 6.000 precari, non potranno neanche amministrare i propri beni perché in luogo della struttura pubblica nascerà una struttura privata che dovrà gestire cinque miliardi l'anno senza nessun controllo pubblico.

In ogni caso, il Partito Democratico - se non si fosse capito - è assolutamente contrario.

**Il Senato non approva.**

Signora Presidente, è vero che Governo e maggioranza hanno finora respinto tutti i nostri emendamenti. Tuttavia, non vogliamo pensare che non ci sia la possibilità di un dialogo, per questo intervengo per sollecitare una particolare attenzione, anche della maggioranza, ad un emendamento che sicuramente può incontrare l'approvazione di tutto il Senato. Con questo emendamento, che propone l'adozione di ricercatori universitari del Mezzogiorno, vogliamo perseguire un duplice obiettivo: da una parte, contrastare la fuga di cervelli dal Sud, che è un gravissimo problema per lo sviluppo del nostro Mezzogiorno e per tutta l'Italia; dall'altra, sostenere progetti di ricerca e di innovazione nelle piccole e medie imprese. Come? Attraverso il meccanismo del credito d'imposta al 60 per cento, per tutti i nuovi contratti stipulati dalle università meridionali per assumere titolari di dottorato di ricerca o laureati. I contratti sono di tre anni e prevedono il cofinanziamento delle Regioni.

Crediamo che ormai il problema sia sufficientemente maturo per essere affrontato in modo definitivo da parte del Senato e, quindi, da parte del Parlamento in quanto sino ad oggi su questo argomento vi è stata molta ipocrisia. Le considerazioni svolte fino ad oggi, se avessero avuto un valore reale, avrebbero dovuto indurre non a mantenere l'attuale quadro dei quattro casinò presenti nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi:

Mi sembra questo un atteggiamento oggettivamente ipocrita che cerca di evitare il problema non affrontando una iniziativa che, tra l'altro, incoraggerebbe maggiormente lo sviluppo turistico del nostro Paese,

consentire al Governo una più attenta riflessione e, quanto meno, rimettersi alle decisioni dell'Assemblea. Non crediamo infatti che questo argomento meriti una considerazione politica di parte,

Il tema delle case da gioco, su cui l'ipocrisia è particolarmente sviluppata in questo Paese, è giunto all'attenzione del Governo in quanto il Ministro per il turismo ha disposto sul tema una proposta massiva,

con una strategia massiva sul nostro territorio attraverso altri meccanismi, diventa scandaloso quando riguarda le case da gioco. Il Mezzogiorno ha pochissimi pochissimi *asset* economici, e quello del turismo viene sempre evocato come una prospettiva di sviluppo importante. Riteniamo che istituire quattro case da gioco nelle Regioni meridionali che hanno vocazione turistica sia giusto e giusto e corretto, quanto meno per parificare l'offerta turistica con il Nord del Paese, che conta quattro case da gioco in località turistiche: Sanremo, Campione d'Italia, Saint Vincent e Venezia. Questa è una proposta minima, dopodiché il tema delle infiltrazioni e del riciclaggio, che ovviamente ci preoccupa, dovrebbe essere superato dalla vigilanza attiva che le autorità di pubblica sicurezza dovrebbero riservare a tali siti, che anzi diventerebbero un luogo privilegiato di verifica dei flussi finanziari. Quindi, come in tutte le altre occasioni in cui investimenti e scelte precise sul Mezzogiorno non possono essere non possono essere operati perché c'è un problema di eventuale infiltrazione malavitosa, basta che lo Stato faccia il proprio dovere e vigili rigorosamente con i suoi organi perché questo pericolo sia escluso. Per tale ragione, se la scelta dei relatori è di chiedere l'accantonamento sono

Ci sono poi queste richieste di accantonamento, che sono ovviamente volte a riconsiderare la situazione per l'eventuale accoglimento degli emendamenti Sono fortemente contrario al fatto che si possano istituire nuovi casinò in Italia, perché i quattro esistenti sono stati stabiliti nel 1927 per ragioni territoriali di frontiera (Sanremo, Campione, Venezia e Saint Vicent), onde evitare che i clienti andassero nelle Nazioni vicine a giocare.

perché quello è un luogo dove si può realizzare il riciclaggio, dove si può recare tutta una serie di persone appartenenti alla malavita

che possono portare criminalità, riciclaggio e soprattutto non devono essere diffusi a livello nazionale, perché faremmo qualcosa di negativo - lo sottolineo - anche sul piano etico.

Le case da gioco non sono la soluzione del turismo italiano. Il problema del turismo italiano è la qualità dell'offerta turistica. *(Applausi dai Gruppi* È necessario sul punto essere chiari, perché non si può parlare di politica turistica in questi termini.

mio terzo tentativo, in questi due giorni, per dire qualcosa all'interno dell'Aula, e non nei corridoi, sulla questione, esplosa sulla stampa e nel chiacchiericcio che ognuno di noi incontra in piazza, al presunto dilagare della droga e degli stupefacenti nel ceto parlamentare. Inoltre, siamo anche destinatari, per un verso, di messaggi, appelli, inviti e sollecitazioni

Essendo tutti noi parlamentari di piazza, di città, di luoghi di lavoro e non di salotto e di triclini, cominciamo ad essere leggermente seccati e anche angosciati da questo tipo di martellamento. Dico chiaramente, gentile signora Presidente, cari colleghi, che fino a pochi giorni fa io avrei ritenuto semplicemente ridicolo, paradossale e offensivo, per me stesso e per altri, avere l'obbligo di sottopormi a un siffatto test, test, al pari di tutti coloro (e voglio sperare che siamo un'ampia maggioranza) che si sono sempre battuti in prima linea per la prevenzione e la repressione del degrado funesto causato

si prenda l'impegno morale di far sì che chi dovesse risultare positivo a questi effetti sia moralmente tenuto a rassegnare le proprie dimissioni. A queste condizioni e alla luce di tali premesse, rassegno l'opportunità alla Presidenza della nostra Camera, che con dignità e coerenza, al di fuori del chiacchiericcio volgare, si prenda una determinazione e la si porti a nostra conoscenza.

suicidi: oltre un terzo. Sono dati al 31 ottobre 2009, che includono Stefano Cucchi ed escludono Giuseppe Saladino, 32 anni, deceduto nel carcere di Parma a meno di ventiquattro ore dall'arresto: stava bene, un malore in cella di notte ed è morto. La procura di Parma ha aperto un'inchiesta. In questi giorni la Commissione di inchiesta sul Servizio sanitario nazionale sta facendo audizioni

L'indagine era nata con lo scopo principale di monitorare lo stato di avanzamento e di passaggio dalla sanità penitenziaria alle ASL e al sistema sanitario nazionale.

associazioni con vari scopi e finalità, alcune con la precisa missione di abolire la caccia. Un accanimento, quello nei confronti della caccia e dei cacciatori una categoria di cittadini onesti che vanta il primato di avere tutti i suoi componenti con la fedina penale pulita, e di questi tempi, signora Presidente, non è poco - portato avanti dalle *lobby* ambientaliste e anticaccia e supportato da gran parte dei media e da alcuni giornalisti del servizio pubblico televisivo. Anche qui avrei qualcosa da dire, visto che gli interventi sono sempre a senso unico contro la caccia, senza mai un contraddittorio, sempre a spese del cittadino. Tutto ciò a fronte della crisi che ha colpito pesantemente l'industria armiera, che nel distretto delle province di Bergamo e Brescia raggiunge l'eccellenza a livello mondiale, e l'indotto, con migliaia di famiglie che si sostentano con l'attività venatoria. Queste industrie, anche a livello artigianale, rappresentano un vanto per il nostro Paese e pertanto vanno sostenute e tutelate. Abbiamo un milione di praticanti, 45.000 addetti al settore e 2.350 milioni di indotto economico.

a finanziarsi e se nei vari capitoli di spesa del bilancio dei Ministeri interessati o nel bilancio generale dello Stato esistano contributi, provvidenze, elargizioni, liberalità o consulenze assegnate a vario titolo alle associazioni Una volta definite l'esistenza e l'entità di tali provvidenze relative agli ultimi quattro anni, chiederò, sulla base dei dati emersi, che sia passata al vaglio da parte delle autorità competenti la congruenza contabile e fiscale nella loro gestione da parte delle associazioni beneficiarie Una di queste - cito, in particolare, la Lega abolizione caccia, come riportato dal suo sito Internet - sta lanciando la notizia che è iniziato l'*iter* del campo antibracconaggio nelle valli bresciane, in collaborazione con un'associazione tedesca. A questi si sono aggiunte decine di volontari giunti da Italia, Germania, Polonia, Gran Bretagna e Stati Uniti, che per tutto il mese di ottobre hanno percorso le valli bresciane, a loro avviso invase da trappole e da reti di cattura. Caratteristiche principali per partecipare a tale corso sono la buona resistenza fisica e la capacità di autocontrollo nelle situazioni di contrasto con i cacciatori.

per malattia e per suicidio, l'amministrazione penitenziaria tiene fermo un concorso già espletato, con le graduatorie già approvate, per quasi 40 psicologi.

Non credo che la vita di un uomo possa essere sottoposta ad un simile condizionamento, ad una folle burocrazia che non consente il superamento di un problema meramente tecnico, cui bisogna fare fronte. Avevo sottoposto questo tema al sottosegretario Caliendo,

banche, derivati e poteri forti. Le banche non danno 100.000 euro ai piccoli imprenditori, ma 800 milioni di euro ai loro amici e sodali. Ieri,

l'articolo, la CONSOB ha esentato le banche dall'obbligo di OPA, per cui di fatto si trovano ad essere gli azionisti di controllo della società, ma non saranno costretti a comprare le quote

con la quale chiedevo al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze di intervenire per fare rispettare dal Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia i contenuti della legge n. 448 del 1998 rispetto ai contributi da dare alle emittenti televisive locali. Questa legge non è stata assolutamente rispettata. Sono stati dati, indebitamente a quanto pare, dei denari ad emittenti televisive, segnatamente una, una, che non aveva assolutamente i requisiti voluti dalla legge. Ho insistito, peraltro, perché la stessa televisione è stata diffidata da RAI Way, che aveva chiesto al Ministro dello sviluppo economico di diffidare l'articolazione periferica del suo Dicastero, e in particolare l'ispettorato territoriale di Calabria, Puglia e Basilicata, a provvedere alla rimozione delle interferenze causate dalla stessa emittente. Tale emittente, peraltro, sentendosi *legibus soluta* ed evidentemente protetta da qualcuno che non intende nemmeno rispondere, continua a fare rispondere, continua a fare trasmissioni decisamente denigratorie nei riguardi della sottoscritta, ma anche di altri soggetti politici che evidentemente non sono graditi ad una parte dei committenti dell'emittente stessa.

senatori Di Giovan Paolo

antidroga. Presenteremo, a questo punto, un'interrogazione parlamentare per avere informazioni in merito. Se poi questi strumenti devono essere utilizzati come liste di proscrizione per l'espulsione dal PdL, è un conto; se invece si vuole addirittura far sospendere qualcuno dalla carica di parlamentare, è un altro. Ricordo che all'interno all'interno della pessima legge Fini-Giovanardi non esiste niente di tutto quello che è stato spiegato dal senatore Benedetti Valentini; sono invece indicate

problemi di costituzionalità da affrontare, rivisitando una legge pessima che ha creato un fenomeno ulteriore rispetto a quello del consumo delle sostanze stupefacenti. Di certo, però, utilizzare ulteriore populismo e demagogia per cercare di affrontare quello che non è un problema - perché qui nessuno fuma

per l'assegnazione della raccolta dei rifiuti speciali ospedalieri. La gara è stata vinta da una società il cui proprietario è tale Ferri e il responsabile dell'ufficio che ha preparato la gara è l'ingegner Ferri.